la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, l'impegno 1) della mozione n. 800 a prima firma del senatore Gotor, per estraneità all'oggetto della discussione.

«Caro Presidente, si fa riferimento alle mozioni parlamentari presentate nei giorni scorsi, con le quali viene richiesto di porre in essere iniziative volte al rinnovo del consiglio di amministrazione della Consip SpA. A tal riguardo appare opportuno informare la Signoria Vostra che l'amministratore delegato ha informato questo Dicastero che sono state presentate, in data 17 giugno 2017, le dimissioni da parte di due consiglieri di amministrazione e che, ai sensi dell'articolo 12.4 dello statuto sociale della Consip, con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione si intende dimissionario l'intero consiglio. L'amministratore delegato, pertanto, sentito il collegio sindacale, ha manifestato l'intendimento di convocare d'urgenza, ai sensi del medesimo statuto, l'assemblea degli azionisti ai fini della ricostituzione del consiglio di amministrazione. La ricostituzione del nuovo organo di amministrazione sarà effettuata secondo le previsioni di legge e di statuto applicabili. Cordiali saluti, Pier Carlo Padoan».

un Parlamento come il nostro, attento anche alla sostanza dei problemi, deve prendere atto il cuore di tutte le mozioni, a cominciare, naturalmente, da quella del senatore Augello, che è stata la prima sull'argomento, ha raggiunto i suoi effetti. effetti. Chiedevamo - l'ha chiesto anche il Partito Democratico con la sua mozione - l'immediata rimozione dei vertici della società

che il consiglio è decaduto. Abbiamo anche appreso - e lo sappiamo - che il giorno 27 del mese corrente, quindi tra una settimana, l'Assemblea è stata convocata per il rinnovo degli organi.

e se tutti noi crediamo alla giustizia, dobbiamo sapere che l'inchiesta deve svolgersi in pace e deve essere seguita con grande rispetto.

che credo sarebbe più utile che questo nostro dibattito si svolgesse dopo il giorno 27 e cioè dopo il rinnovo dei vertici. Ciò ci consentirebbe di discutere sull'attività della società sull'attività della società e quindi sui contenuti. Il Partito Democratico ha preso atto della decadenza del consiglio d'amministrazione ha quindi ritirato la sua mozione iniziale sostituendola con una mozione, con la quale chiede al Governo di procedere al rinnovo del

Fatemi dire, molto banalmente, che il buon senso comune, dal quale anche il Parlamento dovrebbe essere in qualche modo interessato, mi fa interrogare sul senso di un dibattito su una questione già superata e mi fa invece sottolineare che il contenuto di tutte le mozioni,

dalle parole del presidente Grasso, che riferiva della lettera del ministro Padoan.

venga rinviata la discussione delle mozioni? ZANDA *(PD)*. Penso che tutti i presentatori delle mozioni dovrebbero prendere atto del raggiunto risultato richiesto.

Signor Presidente, la lettera del ministro Padoan, che lei ha avuto la cortesia di leggere, pone un problema di carattere formale e un problema di carattere politico. Vengo brevemente al primo aspetto. Bisogna innanzitutto prendere atto del fatto che il ministro Padoan ha cambiato idea: non è la prima volta che gli accade e, d'altra parte, non è nemmeno una cosa sconveniente.

perché sollevi dall'incarico l'ingegner Marroni, si osserva che l'amministratore delegato non si trova in una condizione per la quale lo statuto della società, che ha accolto la direttiva Saccomanni, contempla o prescrive la decadenza». Prendiamo atto che oggi la versione è cambiata. In secondo luogo c'è il problema, dal punto di vista formale, della lettura e della interpretazione dello statuto. dello statuto. Io mi sono applicato a questo esercizio nella giornata di ieri e devo dire che sono arrivato alla conclusione che i vertici Consip dovrebbero essere cacciati quantomeno per il modo in cui lo statuto è stato scritto: è un testo pasticciato e in alcuni punti addirittura surreale. Porto soltanto un esempio. Lo statuto afferma che il consiglio d'amministrazione della Consip è composto da tre membri e, per le diverse procedure da adottare in caso di dimissioni, lo stesso statuto contempla tre ipotesi

sempre di due consiglieri stiamo parlando. Eppure, nel caso di dimissioni della "maggioranza dei consiglieri" e nel caso di dimissioni di "uno o più amministratori" lo statuto prevede due procedure diverse. procedure diverse. Mi sembra che come primo atto bisognerebbe sottoporre lo statuto della Consip ad un accertamento di logica elementare. in uno statuto malscritto vi è un punto comunque inequivocabile, e cioè che il dottor Marroni è al momento assolutamente in carica. A seconda del numero di consiglieri dimissionari lo statuto attribuisce infatti a organismi diversi la prerogativa della convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo degli amministratori: se si dimettono tutti e tre l'assemblea viene convocata dal collegio sindacale, al quale vengono anche demandati nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; se si dimettono due consiglieri, l'assemblea viene convocata dagli amministratori rimasti in carica elemento altrettanto rilevante - a nessun organismo ulteriore vengono demandati gli atti di ordinaria amministrazione. D'altra parte, nella giornata di ieri ha convocato l'assemblea per il 27. Mi sembra quindi evidente che dal punto di vista formale non è possibile sostenere l'avvenuta decadenza, che si perfezionerà nel caso dopo l'assemblea.

fondamentalmente quello di fare chiarezza sui diversi aspetti che si sono condensati attorno alla vicenda Consip. In realtà in quel momento gli aspetti erano due, ma nel frattempo se ne è aggiunto un altro. Da una parte i rapporti oscuri con cordate affaristiche che in qualche modo lambivano la politica, dall'altra un'inchiesta saltata per una fuga di notizie. A questi due aspetti, durante presentazione della mozione, si è aggiunta un'altra vicenda, cioè quella della manomissione della trascrizione di intercettazioni per aggravare la posizione di uno degli indagati.

dal fatto che bisognerebbe affermare quello che in quest'Aula è stato negato, cioè il principio di non contraddizione. Non si può dare ragione nello stesso momento all'accusato e all'accusatore, come a lungo il Governo e la maggioranza hanno preteso di fare. essere rimossa lasciando impregiudicato il giudizio penale, ma rilevando manifeste manifeste violazioni del codice etico, che sono l'aspetto evidenziato dalla nostra mozione e per il quale abbiamo chiesto la revoca dei vertici. In altre parole, signor Presidente, tra Marroni e Lotti noi non abbiamo preso posizione, perché questa è una valutazione che spetta alla magistratura. Semmai, abbiamo sommessamente notato che il ministro Lotti si è comportato in maniera diversa dai suoi predecessori, i quali, sfiorati da dubbi e sospetti, hanno rimesso hanno rimesso il loro mandato. Questa è però una scelta personale del Ministro e non è una cosa che, per quanto ci riguarda e per la nostra coscienza di garantisti, abbiamo chiesto.

per chiedere una discussione pubblica siano aumentate e non diminuite. Quello che è accaduto anche in quest'ultima fase suggerirebbe al Parlamento di svolgere una discussione di questo tipo, anche perché -

che parla della possibilità di revocare le deleghe al ministro Lotti. Allora, se questo è stato

Per quale motivo, a questo punto, far intendere che il Parlamento voglia rimandare o affossare una discussione? Credo che questa discussione si possa affrontare

un dibattito che, invece, anche grazie all'iniziativa parlamentare - e credo anche grazie alla nostra iniziativa - ha fatto dei passi in avanti. Ritengo che il modo migliore per chiudere

il senatore Quagliariello abbia ricostruito con dovizia di particolari gli accadimenti che hanno preceduto gli eventi che anche lei ha citato oggi, leggendo la lettera del ministro Padoan.

come ricordava giustamente il senatore Quagliariello, e ha fatto dare le dimissioni ai due consiglieri che sono di nomina diretta del Ministero dell'economia

agli estensori ed ai firmatari delle mozioni è quella di aggiornare il dispositivo, perché ad esempio il primo punto della mozione a prima firma del senatore Augello sembra essere superato dagli eventi che lei stesso, signor Presidente, in questa sede ha descritto. Al di là di questo, mi pare che tutto rientri nella normalità, nella capacità e nella volontà di questa Assemblea di essere comunque di stimolo e di orientamento per le decisioni che saranno probabilmente prese nella prossima assemblea di Consip.

non è sufficiente a sostanziare la richiesta del presidente Zanda di non procedere alla discussione.

creando, in queste lunghe settimane, da quando è iniziato il tutto, una situazione paradossale: un un amministratore delegato, difeso dal ministro Padoan, che afferma che deve rimanere al suo posto, accusa il

avvenire dandone conto al Parlamento, e cioè secondo i criteri e gli indirizzi della già tanto citata direttiva 24 giugno 2013.

avere un controllo degli appalti, far risparmiare la pubblica amministrazione ed essere, in qualche modo, un argine, con una centrale unica,

di avviare una indagine e una inchiesta amministrativa all'interno della Consip, proprio per verificare tutte le procedure di assegnazione degli appalti. Un'altra questione riguarda la la missione stessa della Consip e, quindi, le modalità e i criteri con cui vengono fatte le gare. Dico questo, signor Presidente, perché - a nostro avviso - le mozioni non possono essere

che va tutto bene, che due vertici su tre si sono dimessi e che l'amministratore delegato - che secondo voi sarebbe azzerato - ha comunque chiesto la convocazione del consiglio di amministrazione. Se uno è azzerato e non c'è più, non chiede la convocazione di niente: al massimo è l'azionista di maggioranza che lo chiede, e cioè il MEF.

l'appalto più grosso di Europa; un imprenditore che si chiama Romeo dà 100.000 euro a un funzionario Consip perché gli interesso una parte di quei 18 lotti la parola «lotti» - e dopo promette dei soldi anche a un altro imprenditore, che si chiama Russo, perché vuole incontrare il padre dell'ex Presidente del Consiglio, nonché

tira in ballo addirittura il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il ministro Lotti, quindi, in questa vicenda non ha una mano nella marmellata: è direttamente nella grande tinozza dove la stanno preparando, vi è dentro fin al collo.

No, assumetevi la responsabilità di discutere, di bocciare le richieste contenute nelle mozioni delle opposizioni ed eventualmente di approvare solamente la vostra. Chiedete agli altri la leale collaborazione di ritirare le mozioni. Ma da quando in qua voi siete stati leali?

per quanto sia necessario e utile nel dibattito tenere conto di quanto avvenuto negli ultimi giorni, le comunicazioni inviateci dal ministro Padoan non appaiono dirimenti per portare alla decadenza o al ritiro delle mozioni. Se è vero che i dispositivi delle diverse mozioni - alla luce della decisione di improponibilità, da parte del Presidente, di uno dei punti della nostra mozione - in parte convergono, le motivazioni che giustificano questi dispositivi, tra cui quella improponibile, restano in piedi. Sono motivazioni anche significativamente diverse tra mozione e mozione: toccano una pluralità di problemi - tra cui lo stretto intreccio tra affari, politica e istituzioni - che vanno oltre alla figura dell'amministratore delegato Marroni e meritano quindi - a nostro avviso - una discussione in questa

la richiesta più volte avanzata che il Presidente del Consiglio valuti la sospensione delle deleghe del ministro per lo sport Luca Lotti, fino al fino al chiarimento della vicenda che lo vede coinvolto, perché il Governo possa operare al riparo da ombre su comportamenti non irreprensibili dei suoi componenti per portare avanti i suoi impegnativi obiettivi.

i lavori parlamentari si sarebbero svolti in siffatto modo. E non voglio entrare nel merito della discussione, che mi auguro potremo affrontare successivamente quando si tratteranno le mozioni. In questa fase preliminare, però, credo che qualche parola vada spesa anche per l'irritualità della discussione che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo vissuto una legislatura nella quale credo sia stato sotto gli occhi di tutti il fatto che il Parlamento, e soprattutto il Senato, sia stato commissariato da un Governo onnipresente. Anche l'irritualità della lettera del ministro Padoan di oggi, che tenta, ancora una volta, di sottrarre il dibattito a un'Aula parlamentare, credo sia un argomento da sottolineare.

relative al rilancio dell'azione della Consip in termini di migliore strutturazione, di trasparenza

Al di là delle considerazioni del senatore Quagliariello, non si può non tenere conto della circostanza che la stessa convocazione dell'amministratore delegato Marroni il giorno 27 è un fatto tecnico consequenziale alla decadenza del consiglio d'amministrazione. quindi, su questo, credo non vi possano essere assolutamente equivoci. Ciò non toglie che si avverte la necessità di discutere della Consip, con suggerimenti

Non ho difficoltà nel riconoscere che, nell'intervento del senatore Zanda, c'è stata l'obiettiva capacità di riconoscere che questa mozione, cento giorni fa, ha aperto una fase di riflessione che ci porta oggi sostanzialmente ad aver allineati sul tavolo documenti che lasciano intendere la possibilità di arrivare a un'indicazione univoca del Parlamento. Dunque, per quali ragioni discuterne comunque e svolgere alcuni necessari approfondimenti attraverso il confronto?

Governo. Oggi stiamo facendo il nostro lavoro e dobbiamo esserne orgogliosi: il Senato della Repubblica sta svolgendo una sua importante attività di indirizzo e controllo rispetto a una situazione, palesemente scappata al controllo del Governo,

dire che soprattutto salta fuori che intorno alla Consip si svolgevano con una certa frequenza colloqui, convegni aperture di credito rispetto a soggetti interessati alle gare che si dovevano svolgere. E lo sappiamo non perché ce lo ha detto un uccellino, ma perché siffatta abitudine - peraltro esplicitamente esclusa, oltre che dal buonsenso, anche dal codice etico della Consip - viene - viene certificata dall'amministratore delegato, ancora oggi in carica, che spiega, anche in alcune interviste, che non soltanto questi colloqui si sono effettivamente svolti, ma che "così fan tutti" e che è *à la page* gestire detto ruolo ascoltando tutti, senza poi truccare le gare. Questo elemento già in sé è un'ottima ragione per aprire una discussione e fare un approfondimento. Com'è stato possibile per cento giorni non assumere alcuna iniziativa rispetto a una situazione che si presentava in questo modo? E soprattutto, colleghi del Partito Democratico,

Non mi importa che qualcuno l'abbia fatto cento giorni fa e qualcun altro dieci ore fa: lo ha fatto il Senato della Repubblica. si deve spiegare perché sia stata necessaria la supplenza; perché - sempre che sia vero, perché nessuno l'ha smentito - sono state respinte per due volte le dimissioni presentate dall'amministratore delegato e per quale oscura ragione soltanto nelle ultime ore vi è stato un cambio di indirizzo. Ripeto che il Senato della Repubblica e i cittadini italiani non lo devono sapere dal Capogruppo del Partito Democratico, che potrebbe tranquillamente risponderci che il Partito Democratico ha presentato la sua mozione alla vigilia del dibattito. È questa, quindi, la posizione del Partito Democratico. Tra l'altro, la prima mozione che presenta il Partito Democratico è, nel *petitum*, sostanzialmente identica alla nostra. La domanda è da porre al Governo ed è il Governo che ci deve una risposta. Questo genere di ripensamenti lascia poi un'altra formidabile

che avevano certo il dovere di informare l'azionista sia di aver saputo che era in corso un'inchiesta, sia di aver deciso di rimuovere le microspie, sia di aver ricevuto pressioni da membri più o meno collegati a forze di maggioranza o, comunque, da persone portatrici di interessi rispetto alle gare? Contrattualmente quei vertici avevano l'obbligo di riferire all'azionista. Perché non l'hanno fatto? Ma, soprattutto, non l'hanno fatto? Queste sono le risposte che deve il Governo e non a noi, che siamo poca cosa, solo dei parlamentari, ma ai cittadini italiani che noi rappresentiamo e che oggi aspettano dal dibattito siffatte risposte. risposte. Ci sono poi altri elementi importanti nella nostra mozione che non riguardano semplicemente l'azzeramento dei vertici della Consip, che ora elenco. Oltre a chiedere risposte, chiediamo che si svolga un approfondimento - come ricordava prima la collega De Petris - a fronte di dichiarazioni di questo genere, riportate dai giornali

Sempre a margine della mozione, perché è importante che noi andiamo fino in fondo oggi e assumiamo delle decisioni, dando questi atti di indirizzo? nelle parole del capogruppo Zanda può essere assoluta, ma, per definizione, non può essere assoluta nei confronti del Governo, specialmente se oggi ci scrive di non preoccuparci perché il consiglio di amministrazione sta comunque decadendo, quando quello stesso Governo aveva respinto le dimissioni dell'amministratore delegato.

di qualche timidezza, signor Presidente. Francamente non so che cosa si agiti nelle scarpe dell'amministratore delegato della Consip. So soltanto che da cento giorni abbiamo una linea molto chiara...

Siamo tutti assolutamente ansiosi di sapere se è vero che l'amministratore ha detto certe cose e quali sono le verità che ci deve rivelare. Non ne abbiamo certo paura e timore e, quindi, vogliamo votare le mozioni, vogliamo dare questo atto di indirizzo e vogliamo essere sicuri che il Governo comprenda che il Parlamento Parlamento vuole esattamente quello che abbiamo scritto nelle mozioni. Signor Presidente, la gente che ci ripensa spesso è imprevedibile e forse è anche meglio per tutti noi, per l'Assemblea e per il futuro della Consip, che la mozione venga illustrata e discussa insieme alle altre, che si approvi un dispositivo e che l'azionista vada

un momento qualificante. In un Parlamento spesso accusato di nascondere o di insabbiare tutto ciò che può creare imbarazzo alla classe politica, il Senato della Repubblica, che è riuscito

una ri-illustrazione, perché già nel mio intervento precedente, nel motivare la necessità di arrivare a una discussione dei testi in esame, ho in qualche modo esposto i motivi di fondo della mozione stessa

per effettuare un controllo sulla spesa pubblica e, quindi, per una razionalizzazione degli acquisti, addirittura con l'ambizione di mettere un freno, grazie a una centrale unica, a un sistema troppo

incappa nella vicenda Consip, nasce da altro. Vorrei ricordare che l'indagine nasce dalla procura antimafia di Napoli su presunti legami con la camorra di alcuni impiegati dell'imprenditore napoletano Romeo e

vorrei qui ricordarlo incidentalmente - anche la Fondazione Open. Andando avanti nel complesso della vicenda, ci troviamo di fronte a una situazione in cui una società interamente pubblica (la Consip) è gestita da un amministratore delegato che

grave perché un Ministro si sarebbe reso responsabile di uno sviamento di indagine ed è attualmente indagato proprio per rilevazione di segreto, per favoreggiamento.

sono un amministratore delegato che accusa un Ministro e un Ministro che respinge l'accusa, ma tutti e due rimangono in carica, e non soltanto perché è stata respinta la mozione di sfiducia il Governo e il Presidente del Consiglio hanno ritenuto di continuare a mantenerlo nella sua carica. Ci troviamo quindi in una situazione kafkiana, che potrebbe avere ulteriori conseguenze.

Come sono state fatte quelle scelte? Con quali criteri sono state scelte quelle persone? Con quali criteri è stato scelto l'amministratore delegato? alle direttive specifiche, da questo punto di vista? Quali erano gli altri *competitor*? Come è stata redatta la *short list*? Tutti questi elementi, che non sono stati osservati, ci dicono esattamente

bisogna assolutamente - questo è l'altro punto per noi assolutamente determinante - ridefinire i criteri delle gare, in modo da consentire non solo la trasparenza, ma anche l'effettiva partecipazione di tutte le imprese, perché è evidente che si era creato un blocco di potere che andava avanti attraverso conoscenze, rapporti e permeabilità della politica, che sono il vero mattone su tutta questa vicenda Consip.

ben espressa dallo stesso presidente Zanda nell'intervento che ha aperto questa sessione. Vorrei davvero che provassimo - cosa che spesso ripetono i colleghi del Movimento 5 Stelle - a spiegare fuori da quest'Aula, ai cittadini che per ventura seguissero questa seduta parlamentare, il senso reale di un dibattito che credo rischi di sfuggire: anche nel combinato disposto fra la lettura dei giornali e quanto il presidente Grasso ha letto rispetto alle comunicazioni del maestro Padoan, questo dibattito sembra surreale. Vorrei sembra surreale. Vorrei che dicessimo ai cittadini - qualcuno lo ha ricordato - cosa è Consip. Consip è quella centrale di acquisto della della pubblica amministrazione che tante volte è stata indicata come uno dei luoghi in cui risolvere uno dei problemi principali di questo Paese, cioè un eccesso di spesa, talora anche scarsamente efficiente. Credo

(la modalità deve ancora essere esplicitata dalla magistratura stessa) risultano coinvolti nell'inchiesta. La novità emersa nelle ultime ore ed in questi giorni e che il presidente Grasso ci ha ben evidenziato, è la lettera del ministro Padoan, esplicitato in quest'Aula quello che abbiamo già letto sulla stampa in questi giorni, e cioè il fatto che i vertici di Consip sono di fatto grazie alle dimissioni di due dei tre componenti del Consiglio di amministrazione e questo ha creato oggettivamente una condizione molto diversa da quella che esisteva che esisteva nel momento in cui sono state presentate le mozioni. Questo è il dato politico e questo è il senso del dibattito di questa mattina ed è questo il motivo per cui è opportuno non continuarlo nei toni con cui era stato anticipato nei giorni precedenti

che il presidente Grasso ha ritenuto inammissibile alla luce di precedenti decisioni già assunte da questa Assemblea, sostanzialmente tutte le mozioni hanno

cosa residua rispetto al dibattito che, oggettivamente, ci ha anche divisi nelle scorse settimane. Qualcuno ha provato a sostenere che l'amministratore Marroni sia oggi ancora in carica: credo bastino nozioni elementari di diritto

fa parte semplicemente degli atti dovuti che gli competono in virtù della sopravvivenza come unico amministratore non dimesso. Credo che questo possa chiudere l'argomento, rispetto a

certi toni di questo dibattito rischino di sminuire tale ruolo, nel momento in cui trasformiamo un tema, che è certamente importante e rispetto al quale vogliamo che la magistratura possa andare fino in fondo, in un dibattito che - mi spiace dirlo ad alcuni colleghi- è è passato da essere un dibattito sostanziale (quello che ancora sopravviveva quando i vertici di Consip erano in carica) a un dibattito meramente formale, con degli accenni

vogliamo venga costruita una strumentale polemica politica su questo tema prima che la magistratura si pronunci.

mai emergere dal dibattito parlamentare nei confronti di un procedimento giudiziario ancora in atto. Inutile ribadire, ma qualche volta è bene farlo, la distinzione dei piani dei poteri è bene primario delle nostre istituzioni. Non vogliamo che, anche in questo caso, si sfrutti questo dibattito per una polemica che possa avvelenare o inquinare la

che questo avvenga nella maniera più trasparente e qualitativa possibile, che le personalità individuate siano del più alto profilo e che (e questo è l'unico

considerato, rispetto ai risultati ottenuti negli ultimi anni, davvero come un patrimonio pubblico da non sprecare. Signora Presidente, onorevoli colleghi, si sarà capito che per Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista la vicenda del Ministro dello sport, Luigi Lotti, e quella dell'amministratore delegato della Consip, dottor Luigi Marroni, sono indissolubilmente intrecciate. È del tutto evidente che uno dei due ha mentito davanti all'autorità giudiziaria e continua a farlo davanti all'opinione pubblica e che la loro contemporanea permanenza in carica, nei rispettivi ruoli, costituisce un inaccettabile segnale di arroganza politica che contribuisce ad aumentare il discredito delle istituzioni pubbliche che abbiamo l'obbligo costituzionale di servire con disciplina e onore. In più occasioni abbiamo sottolineato l'opportunità, se non la necessità, di procedere alla sospensione delle deleghe al ministro dello sport Lotti, fino al chiarimento della vicenda che lo vede coinvolto e continuiamo a ritenere che il Governo debba potere operare al riparo delle ombre su comportamenti non irreprensibili nei suoi componenti per portare avanti i suoi obiettivi. Abbiamo assunto questa decisione a malincuore, essendo una forza della maggioranza di questo Governo, ma siamo stati costretti da un eccesso di reticenza

il dottor Marroni ha prudentemente preferito accettare di fare la parte, tutta manzoniana, del «vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro». Come è noto, nei mesi scorsi, sui principali giornali italiani sono stati pubblicati ampi stralci di dichiarazioni rese in veste di testimone all'autorità giudiziaria il quale ha ribadito gravi affermazioni nei confronti del ministro dello sport Lotti, del presidente Luigi Ferrara, del dottor Filippo Vannoni e di alcuni ufficiali dei Carabinieri, che lo avrebbero informato delle attività investigative messe in atto dalle autorità inquirenti, anche attraverso intercettazioni ambientali negli uffici dei vertici della Consip affinché «le cimici» fossero rimosse, come - questo è il punto - puntualmente è avvenuto. Inoltre, il dottor Luigi Marroni ha dichiarato di avere subìto pressioni per orientare una gara d'appalto indetta dalla Consip da parte del signor Tiziano Renzi (padre dell'*ex* Presidente del Consiglio), il quale è stato anche lui indagato nel medesimo procedimento con l'accusa di concorso in traffico di influenza. Il 9 giugno 2017, in qualità di testimone e, dunque, vincolato all'obbligo della verità, il dottor Luigi Marroni ha confermato la sua versione dei fatti all'autorità giudiziaria e il 17 giugno si sono dimessi dal consiglio di amministrazione della Consip il presidente Luigi Ferrara e la consigliera Maria Oggi chiediamo le dimissioni anche del dottor Marroni, perché ci sembra chiaro che la fuga di notizie relativa all'attività di intercettazione ha oggettivamente ostacolato e messo a rischio il proseguimento di una inchiesta giudiziaria sulla commistione tra politica e affari da quando gli intercettati hanno avuto contezza di esserlo e hanno potuto regolarsi di conseguenza. Nei mesi scorsi abbiamo presentato una mozione di censura specifica, dedicata al ministro Lotti, che attende di essere discussa, con la richiesta di sospendere le deleghe al Ministro dello sport e, in particolare, la delega del CIPE, perché cogliamo un evidente conflitto di interesse tra le competenze della Consip e l'oggetto della delega del CIPE dal momento che, come sappiamo, il ministro Lotti, in qualità di indagato, è comunque all'interno del procedimento giudiziario della vicenda Consip. Occorre prendere atto che quando il dottor Marroni è stato avvisato dell'indagine non ha pensato che fosse suo dovere recarsi immediatamente dalla magistratura per informarla di quanto avvenuto, ma si è affrettato a «bonificare» gli uffici, così da ostacolare il procedimento dell'azione giudiziaria. Tale comportamento appare del tutto inopportuno da parte dell'amministratore delegato di una società a totale partecipazione pubblica, che dovrebbe rispondere, in base allo statuto della Consip stessa, a requisiti improntati alla massima professionalità, onorabilità e correttezza. Tra l'altro, le inchieste giudiziarie di questi mesi riguardanti gli appalti gestiti dalla Consip stanno interessando i vertici e i dirigenti della società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ad esempio come Marco Gasparri, accusato di aver favorito l'imprenditore Alfredo Romeo in cambio di una congrua dazione di denaro, a partire dai bandi del 2012. Questi fatti, purtroppo, fanno pensare che la Consip, nata per centralizzare il controllo della spesa pubblica e attenuare il peso di tante piccole corruzioni locali, abbia di fatto anche centralizzato la corruzione, potenziando il collante tra politica e affari, tra i burocrati che si trasformano in faccendieri e l'amministrazione che diventa un'appendice del politico potente di turno, trascurando qualunque principio di terzietà, efficienza e trasparenza. Fermo restando il sacrosanto principio della presunzione d'innocenza, il punto è che non è necessario attendere che la giustizia faccia il suo corso per rendersi conto di come, nella vicenda Consip, la commistione tra affari e politica abbia dato luogo a un intreccio dannoso per l'autorevolezza e la rispettabilità delle istituzioni. Sarebbe necessario che la politica, in piena autonomia, si autoregolamentasse, elevando l'asticella del rigore e della probità dei comportamenti nella gestione della cosa pubblica e si dotasse di *standard* di condotta omogenei, senza attendere l'intervento della magistratura, così anche da schivare l'apparentemente inevitabile, quanto stantio, dibattito sulla politicizzazione della giustizia, che da troppi anni divide il campo dell'opinione pubblica tra giustizialisti da un lato e garantisti *à la carte* dall'altro. Se la politica agisse prima e con serietà non ingenererebbe il sospetto di una doppia morale e di un garantismo a intermittenza, che trasformano quel principio di civiltà in una mera condotta opportunistica, da rivendicarsi soltanto quando sono coinvolti i propri amici o compagni di partito. la vicenda Consip, a prescindere dal suo eventuale rilievo penale, che spetterà ai giudici valutare, è come una spia dell'olio, che si accende e rivela alcune caratteristiche di fondo del sistema di potere renziano di questi anni, come già la vicenda della Banca Etruria. Anzitutto, il caso Consip ci dice del ruolo del familismo, perché quando si è Presidenti del Consiglio o Ministri *pro tempore,* sarebbe preferibile che i propri genitori si occupassero dei nipoti e non dico sospendessero, ma almeno rallentassero le proprie attività professionali, per evitare di influenzare, con il proprio nome e ruolo, il campo in cui intervengono. In secondo luogo, ci dice anche della messa in pratica di una sorta di chilometro zero del potere, dove tutto si svolge in un fazzoletto di terra in cui si ha l'impressione che il perimetro sia stato troppo spesso tracciato con la squadra e con il compasso toscani. Dico compasso per ricordare agli smemorati che il centrosinistra italiano, nato dall'esperienza dell'Ulivo di Romano Prodi e cresciuto nel PD di Walter Veltroni e Pier Luigi Bersani, aveva a suo fondamento etico-civile la battaglia di Nino Andreatta contro il Banco Ambrosiano, contro Sindona, contro la P2. Oggi quell'esperienza è costretta a mettere nuove radici altrove anche perché è sembrato normale, tranquillo, incontrare - che so io - il faccendiere Flavio Carboni per avere una consulenza bancaria. il caso Consip ci dice delle modalità di finanziamento della politica, delle nuove modalità dopo che, con un madornale errore,

dunque, esercitando un'evidente pressione che già Enrico Berlinguer aveva condannato, ritenendo che la questione morale da affermare fosse proprio quella di un'indebita ed eccessiva sovrapposizione tra ruoli di partito e funzioni pubbliche. E poi ci dice anche dei rapporti finanziari ed economici con il magico mondo del «fu padre costituente Denis Verdini», di cui la politica - e lasciatemelo dire gli equilibri di questo Parlamento, nel corso di passaggi decisivi nell'attuale legislatura sono stati soltanto un vincolante quanto mascherato orpello. Ci dice anche di come una serie di rapporti di origine personale, privatistica e amicale, basati su legami di solidarietà, sono stati predominanti sugli interessi della collettività e sui principi della libera concorrenza e della meritocrazia. Infine, la vicenda Consip, presa nel suo insieme, ci dice del garantismo a intermittenza, inflessibile con gli amici e negato in nome della sensibilità politica e a seguito di pressanti interventi pubblici, nei casi dei ministri Nunzia Di Girolamo, Josefa Idem, Maurizio Lupi e Federica Guidi che furono costretti alle dimissioni. Il punto, tutto politico, è il seguente: ma quale idea di modernizzazione si rivendica e si è proposta in questi anni al nostro Paese? Che tipo di modello imprenditoriale, con quale spazio per la libera concorrenza e la meritocrazia indichiamo all'Italia e ai nostri giovani? Quali rapporti ci sono tra il mondo della politica e quello dell'economia? Ma come è stato possibile, mi chiedo, tradire in modo così manifesto una serie di attese e di speranze che pure c'erano, soltanto in una manciata di anni e nell'arco di un solo giro di giostra nella ruota del potere? Per queste ragioni, Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista chiede di valutare la revoca dell'incarico di amministratore delegato della Consip al dottor Marroni da parte del Ministero dell'economia, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici e la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico. Per questa ragione, Articolo 1 chiede al Presidente del Consiglio di procedere a nuove nomine dei vertici della Consip, seguendo puntualmente e in modo trasparente, e dandone conto al Parlamento, i criteri e gli indirizzi della direttiva a firma del ministro Fabrizio Saccomanni del 24 giugno 2013, che ha rafforzato i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti agli amministratori. È necessario farlo, secondo noi, perché il caso Consip è forse il meno indicato per rivendicare la continuità di questo Esecutivo con quello di Renzi, come ha fatto soltanto pochi giorni fa a Bologna il *premier* Gentiloni, al quale consigliamo di chiudere al più presto questa imbarazzante vicenda nell'interesse del suo Governo, che continuiamo a sostenere, e soprattutto del

Signora Presidente, colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo, oggi, al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. La scorsa settimana, a Busto Arsizio, la mia città, Diana Vrapi Koni è stata uccisa a coltellate dal marito. A lei dedico questo intervento. Ma ancora: A Vergiate, in provincia di Varese, lo scorso 27 maggio, Renata Ottone, di cinquantasette anni, è stata soffocata con un cuscino dal marito, che poi si è suicidato. A Segrate, in provincia di Milano, il 26 maggio, Antonietta di Nunno, una donna di trentacinque anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal proprio *ex*, che si è poi suicidato a sua volta.

ex. Oggi abbiamo anche saputo che la povera ragazza era incinta. Salgono così a 61 le donne che ricordiamo in questo nostro percorso, iniziato solo il 30 giugno 2016. E sarebbero ancora di più se, a Sanremo, due settimane or sono, una ragazzina di tredici anni non fosse riuscita a salvare *in extremis* la propria madre, a cui il padre aveva dato fuoco. I dati presentati dall'ISTAT alla fine di marzo al convegno «La violenza sulle donne: i dati e gli strumenti per la valutazione della violenza di genere» ci dicono che il femminicidio è solo la punta dell'*iceberg* della violenza maschile nei confronti delle donne. In Italia sono oltre 8,3 milioni le donne vittime di violenza psicologica; 4,5 milioni quelle che hanno subìto, nell'arco della propria vita, atti sessuali degradanti e umilianti, rapporti non desiderati e subiti come violenza, abusi o molestie fisiche sessuali gravi, come stupri (653.000) e tentati stupri (746.000).

In una minoranza dei casi, l'l,5 per cento, queste violenze hanno portato a danni seri e permanenti, per strangolamento, ustione o soffocamento. Riproponiamo con convinzione il nostro appello. È un appello al Governo tutto e alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Occorrono risorse, ricerca delle cause, formazione. Occorre un impegno forte. Molte delle donne uccise erano madri o, come nel caso di questa povera donna, lo dovevano diventare. Come è stato stimato dal progetto Switch-off, Switch-off, presentato nei mesi scorsi alla Camera, si stima che nel corso degli ultimi dieci anni siano stati almeno 1.600 i bambini e i ragazzi rimasti orfani di madre o di entrambi i genitori se al femminicidio è seguito il suicidio dell'autore. Un dramma nel dramma. un appello ai *media*: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne, anche quando sembrano difendere i loro carnefici. In un giornale locale in Provincia di Varese è comparso di nuovo l'espressione: «dramma della passione». Non c'è passione se stai a guardare per minuti interminabili, anche venti minuti, una donna che muore perché la strangoli. C'è solo il buio di un orrore indicibile. Un appello al Paese, a uomini e donne: sono state più di 120 le donne uccise nel 2016 e oltre 21 in questo 2017. Tra l'altro, il 2016 è un anno in cui gli altri omicidi sono calati. La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi vogliamo sperare con forza che una società avanzata, civile e democratica non nutra più le cronache di abusi, omicidi e stupri. Non vogliamo, non possiamo più accettare questa mattanza che ci interpella, ci chiama o meglio grida alla nostra coscienza di persone e di legislatori, ogni volta domandandoci se mai finirà questo passaggio di consegne e ogni volta continuandola per non dimenticare, come oggi. *(Applausi

Signora Presidente, nonostante siano alcuni mesi che tento di portare all'attenzione di questa Assemblea le gravi problematiche esistenti nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto e dalle scosse successive, qui non si ottiene alcun risultato. Anche il decreto-legge n. 50 del 2017, che l'Assemblea ha convertito giovedì scorso, è passato senza che il Senato abbia potuto inserire una virgola, eppure quel decreto conteneva circa 15 articoli riferiti al terremoto. I problemi del terremoto sono chiari a tutti: c'è il problema delle risorse, che sono insufficienti e comunque, qualora fossero sufficienti, non vengono erogate al territorio; c'è il problema dell'ampiezza del cratere, che certamente non è adeguata a includere i danni che il terremoto ha procurato nella Regione Marche; ci sono, poi, le norme che rendono praticamente impossibile far fronte all'emergenza e alla ricostruzione. Oggi due giornali di levatura nazionale, quali il «Corriere della sera» e la «Repubblica», si sono accorti di questo stato di cose, quindi non sono

Non solo non si è risolta l'emergenza (perché a febbraio il Governo ha prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza), ma neppure parte la ricostruzione:

nuovo l'inverno e non credo che le popolazioni delle Marche possano affrontare l'inverno nella condizione in cui l'hanno affrontato nell'anno passato. Chiedo che il Senato affronti questo problema, che non può essere risolto

adesso sarà la volta di Errani, perché tra poco gli scade il contratto e non gli verrà rinnovato; poi saranno i Presidenti di Regione a dover rispondere. Ma il dato di fatto è che la condizione delle Marche rispetto al terremoto è quella di partenza. Chiedo che il Senato se ne occupi.

Verona, Brescia e il Trentino. La preoccupazione di tutti noi rappresentanti di queste aree è quella di preservare questo gioiellino, per quello che è dal punto di vista ambientale, ma anche per ciò che rappresenta per le nostre economie.

la rottura di un impianto fognario circumlacuale che è quasi in riva al lago, sul bagnasciuga, poco sotto e a volte affiora. Cosa potrebbe rappresentare? Un danno economico di natura inestimabile, incalcolabile. Il 5 dicembre dell'anno scorso il CIPE ha stanziato finalmente 100 milioni di euro per il rifacimento del sistema fognario del lago, con la condizione che entro un anno si procedesse alla progettazione e alla progettazione esecutiva. La comunità del Garda non ha visto neanche un euro di questi Il progetto complessivamente verrebbe a costare circa 250 milioni di euro: la comunità, le Province e le Regioni faranno la propria parte e i canoni di ammortamento per

e che deve fare tutto il possibile. A questo punto, sia il Governo a comunicare alle amministrazioni locali e alla comunità del Garda questa disponibilità, perché si corra a provvedere a queste opere indispensabili per mantenere questo gioiellino sotto il profilo